sia chiamata a discutere e a votare gli emendamenti riferiti al provvedimento. I tempi sono stati riassegnati in occasione della Conferenza e ovviamente con i lavori di ieri sono stati, in parte, correttamente utilizzati.

Pongo tale questione nel rispetto degli accordi maturati all'interno della Conferenzadei Capigruppo, relativamente sia ai tempi dell'illustrazione e votazione degli emendamenti che all'indicazione della giornata di martedì prossimo per le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento. La questione della inammissibilità concerne il rispetto dell'articolo 97 del nostro Regolamento e dell'articolo 77 della Costituzione. Non mi soffermo in questo momento sul contenuto dell'emendamento, del quale abbiamo già discusso ieri con riferimento agli aspetti di rottura della legalità costituzionale. Segnalo, peraltro, con richiamo al nostro Regolamento, in particolare ad una decisione del 1984 della Giunta per il Regolamento, che i presupposti concernenti gli emendamenti devono essere valutati con particolare rigore. Diceva quel parere "in modo particolarmente rigoroso" in ordine sia ai presupposti di estraneità all'oggetto della discussione, sia in relazione ai caratteri di necessità e urgenza che deve rivestire il nuovo emendamento che in questo caso è stato proposto dal Governo.

al Presidente del Senato - debbano essere distrutti, c'è una corrispondenza tra questo emendamento e l'articolo 2; in altri casi, non c'è assolutamente corrispondenza. Quindi, la questione di ammissibilità viene posta sia sui requisiti di urgenza e necessità, sia in relazione all'estraneità dell'emendamento all'insieme dell'articolo 2.

Grazie Presidente, vorrei chiederle l'applicazione del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, relativamente al noto emendamento di cui stiamo discutendo. Come lei ben sa, questa norma regolamentare prevede che «nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti». Non occorrono argomenti oltre aquelli già ampiamente spesi nella discussione di ieri e a quelli già utilizzati dai colleghi che mi hanno preceduto per motivare un'istanza di tal genere. Al di là del Al di là del gravissimo *vulnus* costituzionale che la norma proposta produrrebbe per le ragioni che sono state - ripeto - ampiamente illustrate, è difficile negare che vi sia la necessità di una valutazione approfondita, di merito di una norma che è molto più complessa di quanto si possa apprezzare da una prima lettura sommaria. Basta Basta riflettere, signor Presidente, sul fatto che la portata della norma si riferisce a tutti i processi e non solo a quelli fissati da qui ad un anno, cioè dall'entrata in vigore della legge ad un anno. Essa si riferisce a tutti i processi individuati nel comma 1

sia sulle parti civili costituite nei processi sia sugli imputati, magari quelli che da anni attendono di ottenere una pronuncia di assoluzione.

Collega Legnini, purtroppo non è così. La Conferenza dei Capigruppo è stata chiara e ha previsto che nella giornata di oggi, entro le ore 20,30, l'Aula esiti le illustrazioni e i voti su tutti gli emendamenti.

questo è il momento in cui possono essere sollevate le questioni di inammissibilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento. Mirichiamo all'intervento del senatore Casson abusando anch'io della lettura del precedente che sul caso specifico ha visto la pronuncia della Giunta per il Regolamento, ossia l'affermazione del principio che nel momento in cui si esamina un decreto assistito dall'urgenza prevista dall'articolo 77 della Costituzione debba esserci la garanzia per un tragitto che non consenta di far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dall'urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

che tenga conto anche dell'indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78». Richiamo ora il preambolo del decreto-legge firmato dal Presidente della Repubblica, che recita come segue: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati alla immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime».

ed *e)* dell'articolo 1 vengono introdotte alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». «L'inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie

ieri abbiamo approvato alcune norme che inaspriscono le pene per queste condotte criminose, per le quali si è ritenuto di intervenire con decretazione d'urgenza. Ieri abbiamo aggravato le pene per il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ma è mai pensabile che nel medesimo decreto che affronta questo tema, inasprendo le sanzioni, sia contenuta un'altra norma che sospende i processi per l'omicidio colposo per oltre un anno? Mi chiedo dove sia la coerenza del decreto d'urgenza se, da una parte, si inaspriscono le pene e si ritiene che si debba intervenire con risposte urgenti rispetto a fenomeni allarmanti e, dall'altra, si inserisce con decretazione d'urgenza la sospensione per un anno ed oltre degli stessi processi. Quello al nostro esame è un decreto incoerente e schizofrenico, perché afferma con decretazione d'urgenza due principi contrari e contrastanti! Non vi è armonia.

previsioni sanzionatorie. Allora, rispetto a questo conflitto logico, giuridico

ai cittadini dobbiamo dare risposte chiare e non risposte equivoche e strabiche, perché questo è ciò che stiamo facendo.

La Presidenza ha valutato attentamente l'emendamento 2.0.800 dei relatori ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento circa l'attinenza all'oggetto della discussione e alla luce del parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984. Coerentemente con le premesse al decreto-legge, relative alla necessità e urgenza «di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa», lo scopo dell'emendamento richiamato - insieme agli emendamenti 2.0.801 dei relatori e 2.0.900 del Governo, sulla precedenza assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza ai delitti più gravi e a quelli commessi in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, con cui si pone in stretta connessione - è quello di concentrare la repressione penale anzitutto sui reati più gravi, puniti con pene più severe, ma anche su quelli avvertiti in modo più sensibile dall'opinione pubblica e tali da suscitare forte allarme sociale. Su tali presupposti, la Presidenza ritiene ammissibile, conformemente all'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento in questione sia sotto il profilo della attinenza per materia - giacché il decreto-legge contiene numerose disposizioni in materia processuale penale sia sotto il profilo delle finalità del decreto medesimo richiamate dal Governo nelle premesse al provvedimento, anche con riguardo ai requisiti di necessità e urgenza connessi alla estrema sensibilità da tutti avvertita su questi temi. Infine, la Presidenza non può non tenere conto, pur nel quadro delle recenti pronunce della Corte costituzionale, di quella che è la prassi costante del Senato, consolidatasi nelle decisioni assunte dalle Presidenze che si sono avvicendate nel corso degli anni precedenti.

la Commissione affari costituzionali, diversamente dalla 5a Commissione, non è interlocutrice diretta per i pareri sui provvedimenti di legge e quindi sugli eventuali profili

la richiesta del senatore Legnini, mi sono permesso poc'anzi di ricordare al collega Legnini il contenuto della Conferenza dei Capigruppo e, proprio in sintonia con quella intesa, ormai la Presidenza ritiene inopportuno un arresto dei lavori dell'Assemblea anche perché, ripeto, il dibattito è avviato e credo che tutti i colleghi siano ampiamente informati

anche per sottolineare che con quell'intesa sarebbe assolutamente compatibile un rinvio anche molto breve, in mattinata, del provvedimento in Commissione,

lettera dava come principale ed evidente motivazione di quell'emendamento la necessità di sospendere un processo a carico del Presidente del Consiglio per dargli il tempo di approvare una legge che escludesse in modo perpetuo

Vivaddio! Vogliamo capire perché lo stesso metro non viene usato per analoghe e ben più gravi norme introdotte in sede di conversione del decreto-legge al nostro esame. Tant'è, ne prendiamo atto e vogliamo che a verbale risultino i due pesi e le due misure con cui il Governo si sta muovendo in una delicatissima materia:

Se fosse questo il vero motivo probabilmente con un po' di buona volontà riusciremmo in questa sede ad approvare una norma più appropriata.

alla legislazione che si vuole introdurre, sbagliata dal punto di vista

di consegnare al Paese dei testi comprensibili, rispettosi delle leggi esistenti esistenti e dei criteri generali del nostro ordinamento giuridico. Gli emendamenti

introducono una modifica dell'articolo 132‑*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

incidere sui poteri discrezionali dei capi degli uffici introducendo un principio ed un criterio di tassatività.

sui poteri di discrezionalità dei capi degli uffici per stabilire in forma tassativa quali siano quali siano i processi che debbano essere celebrati prima degli altri. Strettamente correlato all'emendamento 2.0.801, che modifica l'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, è l'emendamento 2.0.800,

per fatti commessi entro il 30 giugno 2002 anche qualora tali processi si trovino in fase di discussione, ossia abbiano già visto la luce della possibile fine. Si dice, infatti, nessun potere discrezionale, che tutti questi processi devono essere immediatamente sospesi per un anno. Stiamo parlando di rapina, di estorsione, di furto in abitazione, di furto con strappo, di omicidio colposo, di sfruttamento della prostituzione minorile, della violenza sessuale, del sequestro di persona, della calunnia, della subornazione di testimoni, del favoreggiamento reale, dell'incendio doloso, della detenzione di esplosivo a fine di attentato, del falso in atto pubblico, della diffusione dolosa di malattie, delle frodi contro le industrie nazionali, dei maltrattamenti in famiglia contro minori, della circonvenzione di persone incapaci, della frode in emigrazione, della ricettazione, dell'illecita concorrenza con violenza o minacce: vi ho citato solo i più significativi processi che riguardano questi fatti e per i quali si impone la sospensione per legge. Si dice che comunque la sospensione comporta il congelamento dello scorrere dei tempi di prescrizione: è un inganno, e voi lo sapete, perché la sospensione del decorso della prescrizione dura quanto la sospensione del processo indicata dalla legge, ossia un anno, ma poi i termini, cessato l'anno, ricominciano a decorrere fino a quando il processo non verrà rifissato. Quindi, questa norma incide sulla prescrizione.

bisognerà ricominciare da capo, con i termini di prescrizione che continuano a decorrere. Questa è una norma finalizzata a far prescrivere i processi, perché la sospensione che voi introducete è di un anno ma i termini sono molto più ampi. Ma quale tolleranza zero? Quale tolleranza zero? con un sacrificio enorme per le vittime. La vittima di un reato che si sia costituita parte civile e che veda la possibilità di conclusione del processo, giunto nella fase di discussione, si vede improvvisamente sospeso il processo,

e in quella sede, con una norma che voi volete introdurre, l'imputato potrà alzarsi e chiedere il patteggiamento, perché vengono riaperti i termini del patteggiamento; in tal modo, la vittima di un reato che finalmente è arrivata alla fase di discussione del processo che l'ha vista, appunto, vittima attenderà due anni e poi l'imputato chiederà il patteggiamento e la vittima dovrà ricominciare da capo. Questa non è tolleranza zero, questo significa venire incontro ai delinquenti contro le vittime dei reati. Vi è poi un altro inganno che state perpetrando:

danneggiata dalla sospensione del processo di cui vede già la conclusione potrà trasferire l'azione in sede civile. Questa è una cosa che già esiste nel nostro codice, non state concedendo un bel nulla,

che inizia perché la parte civile trasferisce la sua domanda in quella sede dovrà essere sospeso sin quando non diventerà definitiva la sentenza penale di un processo che invece è stato sospeso per legge. Questo è un imbroglio

che il Presidente del tribunale può sospendere i processi qualora i reati per cui si procede siano prossimi alla prescrizione e la pena sia indultabile; non si dice però per quanto tempo: avete scritto una norma per cui un magistrato può sospendere un processo e non si sa per quanto tempo. È un assurdo questo,

questa? Secondo voi, è irrilevante il diritto che può conseguire una parte civile da un'affermazione di responsabilità, anche se la pena è indultabile? L'indulto riguarda le condanne e presuppone l'affermazione di responsabilità: non è indifferente per la parte civile avere una pronunzia di questo tipo, anche se la condanna è indultata, perché la sentenza comunque è affermativa di responsabilità; voi questi processi prevedete che possano essere sospesi per sempre, perché non vi è una scadenza.

quelli che possono essere celebrati devono andare avanti, quale è la terza categoria di processi per i quali la sospensione da obbligatoria diventa facoltativa? A quali processi intendete riferirvi? I presentatori dovrebbero avere il dovere di dare risposta alla domanda su questi altri processi, siano quelli per i quali è obbligatoria la celebrazione prioritaria. Voi, infatti, inserite una terza categoria di processi incomprensibile. è poi questa presa in giro della richiesta di patteggiamento che deve proporsi entro tre giorni dalla sospensione *ope legis* (che scatta, cioè, immediatamente con l'entrata in vigore del decreto) oppure oppure che può proporsi alla prima udienza utile, laddove la prima udienza utile di un processo sospeso si avrà quando il processo verrà rifissato (ossia dopo due anni di attesa). Ora, tutto ciò è assolutamente incomprensibile. In nome di cosa si chiede il sacrificio di migliaia e migliaia di cittadini, di decine di migliaia di cittadini che attendono l'esito di un processo? In nome di cosa si chiede questo sacrificio? In nome di cosa,

Solo per chi non vuole il processo vi è coincidenza di interessi! Non c'entrano i cittadini, che sono danneggiati da questa paralisi che si vuole introdurre nel nostro sistema. Questa non è una risposta di giustizia. Appellatevi alle vostre coscienze e rispondetemi col codice alla mano, se avete argomenti; contestate almeno uno degli argomenti che ho indicato; ditemi quale di questi argomenti è errato, ma fatelo con il codice alla mano! mano! Se non lo fate, questo non è più il Parlamento ma diventa la sede di ratifica dei voleri del principe e non è più il Parlamento!

Sento dire dal Governo che non si possono immediatamente fare norme che impedirebbero la morte di tante persone: io mi auguro che non succeda, mi auguro che non accada un altro caso di *stalking* seguito da morte,

chiedo che almeno sulle misure che riguardano le vittime, il risarcimento del danno che condiziona la sospensione condizionale della pena, la possibilità di fare un incidente probatorio protetto, la possibilità di intervenire, quindi, a favore delle vittime,

quindi, di questo emendamento va in quella direzione ed è per questo che il Governo chiede di modificare la norma votata in Commissione. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 2.0.801;

muovono dal fatto che il sistema penale risulta al collasso - uso frasi non mie. Si è parlato di aggravamento della crisi della giustizia, di perdita di credibilità del sistema giudiziario, di una drammatica crisi di effettività del sistema della giustizia penale, di gravissima crisi di efficienza e funzionalità; si è infine detto che il problema centrale della giustizia è quello della durata dei processi. L'emendamento 2.0.801

questa scelta viene effettuata, giacché nel decreto legislativo riguardante le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado era stato asserito che, al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella della discussione del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che ne può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti.

diede conto della delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura il 15 maggio 2007 aveva preso atto dell'adeguatezza dei modelli organizzativi adottati con la circolare del procuratore Maddalena, ne condivise e difese l'operato al punto da concludere che venivano offerte soluzioni realistiche, razionali, controllabili e complessivamente compatibili con il principio costituzionale di obbligatorietà Per questi motivi abbiamo ritenuto di dover presentare questo emendamento

penale, così come lo sono stati tutti coloro che si sono occupati di questa materia sino ad oggi, anche con qualche caduta di stile. Ho una grande stima per una persona che è stata Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato e che oggi è Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura il quale, con tono perentorio, oggi riferisce a un grande quotidiano che la Consulta dirà che questa norma è incostituzionale. Non credo che il compito di un Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura sia prevedere prevedere tassativamente attraverso gli organi di stampa quello che la Consulta dovrà fare o meno. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Egli è libero di esprimere una propria opinione, ma non di dettare attraverso interviste alla stampa comportamenti ad un organo della cui autonomia credo dobbiamo essere

Signor Presidente, sia nella giornata di ieri che questa mattina i colleghi dell'opposizione hanno abbondantemente illustrato

dovrà essere messo in votazione successivamente, e non prima, dell'emendamento 2.0.801 perché non ne è la premessa, bensì la logica conseguenza.

con tutta una serie di reati per i quali si creano delle corsie preferenziali. Un autorevolissimo senatore dell'opposizione, già magistrato, in occasione

prevede una corsia preferenziale soltanto per i procedimenti in cui vi sono imputati detenuti con scadenza del termine di custodia cautelare. Quindi,

vi è più di un dubbio di ritenere che questi processi vengano avviati in funzione delle idee politiche degli imputati e degli indagati, a discapito di altri procedimenti per i quali non si procede e li si tiene nel cassetto. Il senatore Li Gotti ha scrupolosamente indicato i reati per i quali non ci sarebbe questa corsia preferenziale e nell'emendamento successivo non ci sarebbe poi la sospensione dei procedimenti per un anno. A tale riguardo, voglio ricordare al senatore Li Gotti

non sono soltanto quelli che prevedono disposizioni contro la criminalità organizzata o per i quali la pena edittale massima è superiore a dieci anni.

e quelli, per converso, che non devono essere sospesi stante la gravità dei reati medesimi e l'allarme sociale che suscitano presso la collettività.

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; associazione di tipo mafioso; sequestro di persone a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; ricostituzione di associazioni sovversive; partecipazione a banda armata; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di di armi da guerra o di tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenni; violenza sessuale di gruppo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo vi sia alcun senatore della Repubblica che possa dubitare della assoluta gravità di tali reati e dell'enorme allarme sociale che questi suscitano presso l'opinione pubblica.

Il senatore Vizzini ha riferito quanto è sotto gli occhi di tutti, vale a dire il collasso della giustizia civile e, per quanto ci riguarda oggi, della giustizia penale. Cercare di agevolare la trattazione dei processi per i reati più gravi e che destano maggiore allarme sociale è un'esigenza sentita non soltanto in questo Parlamento, ma presso l'opinione pubblica. l'opinione pubblica. Noi non possiamo non prendere in considerazione l'opinione pubblica: c'è chi sostiene che le elezioni siano state decise proprio sulla questione della sicurezza;

uno Stato debba garantire la celebrazione dei processi per i reati più gravi e, per fare questo, non può che sospendere per un anno la celebrazione dei processi relativi ad altri reati che - ripeto

perché diversamente, onorevoli colleghi, non ci si deve meravigliare...

Siamo tenuti a preconfezionare delle leggi astrattamente valide per tutti. Non possiamo predisporre leggi che valgono per tutti eccettuato qualcuno.

Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore

in relazione alle corsie privilegiate dei processi penali, non è di oggi. Ricordo che il Consiglio superiore della magistratura,

a dare una indicazione ben precisa con circolare sui procedimenti penali che dovevano essere trattati con precedenza. Successivamente abbiamo ricevuto una serie di indicazioni dai procuratori della Repubblica attraverso varie circolari che fissavano criteri di priorità nella trattazione dei processi. Il dibattito culturale e politico, al contrario, era concentrato sulla necessità che fosse il Parlamento

proprio per salvare il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la circolare del procuratore della Repubblica porta ad una sospensione di fatto degli altri processi

Rispetto a questa situazione il Parlamento, con la normativa riguardante il giudice unico, nel 1998 indicato una serie di criteri prioritari da seguire nella celebrazione dei processi. Pur avendo fatto il magistrato per tutta la vita, reputo corretto

garantire che tutti i processi possano essere svolti e celebrati secondo termini e tempi della ragionevole durata del processo.

Se così non fosse, ossia se non fosse prevista la sospensione della prescrizione, avremo né più né meno l'effetto di determinare la caducazione di quelle indagini e di quei procedimenti che il Governo non intende abbandonare. Per tale ragione, esprimo parere favorevole sui due emendamenti

tecnico- funzionale di grande rilievo, che ho cercato di spiegare in sede di Commissioni riunite e che, al di là della ragione datami per le vie brevi, non vedo come affermare se non prendendo la parola.

modifica ha lo scopo di evitare che i magistrati della procura della Repubblica del capoluogo di distretto si debbano spostare per recarsi ai tribunali compresi nel loro distretto

bisogna andare tutti a Torino perché un sostituto procuratore non può andare a tenere un'udienza presso il tribunale di Novara o di Alessandria o di dove preferite. Potrei portare esempi di altri 136 tribunali d'Italia. Premesso che questo non è un profilo ideologico, ma tecnico-funzionale di primario rilievo e premesso che abbiamo sempre sostenuto che è male che ci sia una estrema domestichezza o dimestichezza tra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari,

senatore D'Ambrosio)*. Illustre collega, lei potrà prendere la parola e replicare. Sto sostenendo che stiamo venendo incontro solamente alle esigenze egoistiche dei magistrati delle procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e forse anche, e lo dico, degli studi legali monopolisti dei grandi centri, che accorpano naturalmente le attività giudiziarie di difesa e di supporto, e stiamo realizzando un'opera che ideologicamente non è giustificata da

di sedentarietà di un ristrettissimo numero di magistrati compromettiamo l'attività di molti magistrati e avvocati delle parti e delle realtà giudiziarie

Nessuna scelta di comodità per nessun singolo sostituto procuratore o singolo giudice, ma una scelta di funzionalità perfettamente conforme ai principi del giudice naturale sanciti dalla Costituzione; così come è conforme la disciplina delle Direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale antimafia, con corrispondenti Gip e Gup, varata nel 1992, che qualche risultato ha prodotto. Stiamo qui parlando di terrorismo. Da anni si discute, nelle sedi più appropriate, della inopportunità che il giudice di un tribunale periferico, che fa mille cose durante la giornata, tratti materie che richiedono una specializzazione, di fatto e di diritto, che, come avviene per il contrasto alla criminalità organizzata, non può non esserci per il contrasto al terrorismo,

parere contrario.

*(PdL)*. Signor Presidente, siamo al secondo capitolo dell'argomento sul quale vi ho intrattenuto prima. Naturalmente faccio ossequio alla volontà del Senato,

2.100 che stiamo mettendo ora in votazione. Mi sembra ci sia una incompatibilità, nel senso che, una volta recepito il pur sbagliato

voglio cortesemente rispondere alla persona che forse su questo argomento più stimo, che è Alfredo Mantovano, al quale voglio anche bene: non è affatto vero che ci stiamo occupando solo di terrorismo, ma di tutta quella serie di reati che prima il senatore Berselli ha elencato, che vanno dalla prostituzione alla droga, all'informatica, e via dicendo. Quindi, stiamo spogliando le sedi giudiziarie italiane di una parte importante, quantitativa e qualitativa, della loro competenza come giudice naturale: questo stiamo facendo, cerchiamo di capirci, altrimenti non saremmo neppure avvocatucci di provincia, avremmo fatto un errore da scuola elementare. Così al limite non è, mi meraviglio che i proponenti sostanziali di questa norma, che sono i magistrati del Gruppo PD, anche nelle nostre Commissioni, abbiano ribattuto solo con dei "no" apodittici agli argomenti credo non privi di

quindi di non insistere nell'errore, anche perché con l'emendamento 2.100 andremmo a sovrapporre un secondo errore funzionale a quello che già abbiamo licenziato, con profili di incompatibilità.

Signor Presidente, le chiedo solo un po' più di attenzione quando alziamo la mano, per non dover sbraitare in quest'Aula così aulica.

che il testo che stiamo per a votare, che è un emendamento al famoso emendamento del Governo che chiede di sospendere i processi penali relativi ai fatti commessi fino al 30 giugno 2002, fino al 30 giugno 2002, vada approvato. I relatori, sia il relatore Berselli, sia il relatore Vizzini, sia il Governo hanno cercato di spiegarci e di convincerci che l'intento di questo provvedimento sarebbe quello di privilegiare alcuni processi per reati di particolare disvalore sociale e ci hanno detto che la giustizia è al collasso e quindi dobbiamo procedere con questa modalità.

A parte che è evidente che in una fase di transizione, quindi con l'istituzione di una nuova figura giurisdizionale, può essere giustificato che siano indicati dei criteri prioritari di trattazione, ma poi vorrei ricordare - lo ha detto lo stesso relatore Vizzini - che in quel provvedimento si diceva testualmente: «indipendentemente dalla data di commissione del reato». Nel provvedimento che il Governo propone, invece, abbiamo la sospensione dei processi per i reati commessi fino al 30 giugno 2002: è evidente che le giustificazioni che i relatori vogliono darci, utilizzando come termine di paragone il provvedimento sul giudice unico, questo *vulnus* gravissimo, visto che nella normativa sul giudice unico non era previsto un limite temporale di commissione dei reati; invece qui combinazione, il Governo né i relatori ci hanno spiegato come mai è stato individuato come termine proprio il 30 giungo 2002) abbiamo un limite temporale che a mio parere, essendo io anche un avvocato, è assolutamente ingiustificato.

dalle argomentazioni fra il politico e il giuridico che lei utilizzava per sostenere questo provvedimento e devo dire che sono rimasta tanto più

soggetto che frequenta le aule di giustizia. Quindi, affermare che questi provvedimenti servono per rendere giustizia e accelerare processi aventi particolare disvalore sociale, vuol dire

che ci saranno (come ricordava ieri il collega Morando), rappresentano un problema vero e concreto che metterà in grossa difficoltà i nostri uffici giudiziari. Concludo riportando un'altra citazione, che ho trascritto per non sbagliare, fatta sempre dal collega Berselli. Lei ha detto che non possiamo fare leggi che valgono per qualcuno e non per tutti. Io le dico anche che non possiamo fare leggi che valgano per una persona sola!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi non parteciperemo alla votazione di questo emendamento e ancora ribadisco, se vi fosse una possibilità, che qualora voi ritiraste l'emendamento potremmo tornare a discuterne il merito. Ma è esattamente il merito quello che non viene in discussione in quest'Aula e che non è venuto in discussione in Commissione, che non si è occupata

Governo e delle Commissioni. Nessun argomento di merito tranne quello, simbolico ma menzognero, per cui questa è una norma che servirebbe per aumentare le condizioni di sicurezza nel Paese, consentendo ai cittadini di vedere celebrati subito i processi per i fatti più recenti e impressivi, lasciando fuori di giustizia non soltanto le ragioni di quegli imputati, anche innocenti (molto innocenti) che sono sotto processo e che vedono sospeso il diritto a vedere proclamata la propria innocenza, ma anche - come ci ha illustrato il senatore Li Gotti - di quelle parti civili che per troppi anni hanno atteso giustizia. E questo riguarda anche processi molto seri, per fatti molto gravi: ne cito soltanto uno, quello che riguarda i fatti di Bolzaneto. Nessun argomento di merito, dunque. Io, invece, vorrei aggiungere qualche argomento di merito per giustificare la nostra posizione, che non è pregiudiziale, non è figlia dell'antiberlusconismo, (la voglio dire, questa cosa, la voglio dire chiaramente) dire chiaramente) ma nasce dall'esperienza di chiunque abbia frequentato le aule di giustizia, e ce ne sono tantissimi di autorevoli tra i vostri banchi. Sapete benissimo

di inviare a tutte le parti del processo la comunicazione della sospensione. E questo ovviamente non riempirà automaticamente i ruoli del processo, perché questi si preparano con largo anticipo e voi sapete quanto tempo occorre per le notifiche, per le notifiche, perché vadano a buon fine e siano rispettati i termini del processo. Noi avremo un pezzo del lavoro dei nostri tribunali che sarà non utilizzato: altro che contributo alla sicurezza!

non è una sofisticheria ideologica. Voglio dirlo con chiarezza, perché credo davvero che dirci le cose così come le pensiamo possa essere il modo migliore per venir fuori anche da momenti aspri e difficili di conflitto come questi. Il senatore Zanda poco fa ha adoperato un argomento per contestare, ovviamente in piena legittimità e senza nessun attentato all'autorità del Presidente del Senato, la sua decisione secondo la quale l'emendamento viene ammesso perché è coerente con i fini del decreto-legge, che è quello di raggiungere un maggior livello di sicurezza; e lo ha fatto partendo dalla lettera del Presidente del Consiglio. Colleghi, la logica non è a disposizione di una parte, ma è - come dire - il presupposto stesso della capacità di intendersi: quando il Presidente del Consiglio, anche con un certo allarme, segnala nella propria lettera che i suoi legali lo hanno informato che tra i processi che verrebbero sospesi (stendo un velo pietoso su tutto il resto) ci sarebbe anche il proprio, la logica avrebbe voluto che il presidente Berlusconi annunciasse al Presidente del Senato il ritiro dell'emendamento e non il fatto che avrebbe presentato un disegno di legge sull'immunità per le alte cariche dello Stato! *(Applausi dal

Forse il presidente Berlusconi con questa norma e poi con la misura sull'immunità per le alte cariche dello Stato sfuggirà a una sentenza, peraltro di primo grado, ma perderà una grande

l'uscita dalla transizione italiana e l'inizio di una nuova era del bipolarismo in Italia, in uno schema politico semplificato grazie a noi e nella possibilità vera di ridare forza alla democrazia italiana. sta sprecando un'occasione e la state sprecando anche voi. Torneremo a vedere un film già visto, coronato ancora una volta dall'intervento della Corte costituzionale. Non è questa la politica che mi sarebbe piaciuto vedere. *(Vivi,

La prima questione riguarda il fatto che si interviene sull'articolo 132*-bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stravolgendone natura e finalità. Il testo originario prevede infatti una valutazione di sostanziale parità per tutti i processi e per qualunque reato, tutti considerati su un piano paritario ad eccezione di quelli con imputati in custodia cautelare,

Solo questa esigenza, connessa ad un'urgenza temporale, determina la preferenza per tali procedimenti. La nuova regola, invece, svilisce tale criterio; non si fa più alcun riferimento alla prossima scadenza delle misure cautelari, anzi, al contrario, dà preferenza a procedimenti per reati che hanno i più lunghi termini di prescrizione rispetto a procedimenti per reati meno gravi che si prescrivono più velocemente. Il risultato pratico sarà la verosimile prescrizione di moltissimi procedimenti per reati solo formalmente meno gravi di quelli indicati. Si pensi alla casistica già citata, alla quale mi permetto di aggiungere qualche altra ipotesi di reato quali: il peculato e la malversazione ai danni dello Stato, la corruzione e la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione, l'abuso d'ufficio, la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, la calunnia e l'autocalunnia, le false informazioni al pubblico ministero, la falsa testimonianza e la subornazione di testimoni, favoreggiamento reale e personale, l'incendio e l'incendio boschivo e quant'altro. La lista è lunga. Ad esempio, da ultimo, i reati in materia ambientale e di gestione e traffico illecito di rifiuti. Ovviamente, una scelta di tale genere si pone evidentemente in contrasto con altre norme del cosiddetto pacchetto sicurezza che, invece, aumenta le pene per gli omicidi colposi da incidenti stradali, modifica le regole di giurisdizione e di controllo del territorio in materia di rifiuti, cerca di prevedere regole che diano maggiore sicurezza al cittadino nella vita di tutti i giorni. Ma poi stabilisce che i processi per fatti di questo tipo non debbano essere celebrati (ovvero possano esserlo solo dopo altri). La norma dell'articolo 132-*bis*,così come modificata dai citati emendamenti, appare poi in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione sull'obbligatorietà dell'azione penale. Tale principio non riguarda solo la condotta del pubblico ministero; non impone, cioè, solo al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, ma sta a significare che l'intera organizzazione giudiziaria statale deve perseguire tutti i reati, senza distinzione.

Con la conseguenza che un procedimento con imputati con misura cautelare in scadenza ben potrebbe essere ritardato per trattare nei ruoli d'udienza altri procedimenti indicati dalla norma emendata, non esistendo alcun ordine di preferenza né alcuna regola di priorità, se non quella del buon senso del giudice del caso concreto. Altra anomalia della norma nel testo derivante dagli emendamenti è che verrebbe data priorità assoluta a procedimenti per reati - quelli commessi in violazione della normativa antinfortunistica - che ovviamente importanti in ottica sociale ed in un momento in cui le morti bianche riempiono le cronache, si risolvono però spesso in procedimenti per contravvenzioni bagatellari

ma fa riferimento generico ai reati di tale tipo. E statisticamente la maggior parte dei reati riguarda reati contravvenzionali puniti in maniera irrisoria. La conseguenza potrebbe essere la seguente: che un processo per usura o per omicidio colposo da incidente stradale dovrebbe lasciare il passo ad un processo per una contravvenzione per non aver esposto i prescritti cartelli nel cantiere o per aver fornito all'operaio una scala non in regola. Appare poi francamente incomprensibile, signor Presidente, il riferimento, come elemento che attribuisce al procedimento priorità assoluta sugli altri, al fatto che l'imputato sia detenuto anche per reato diverso da quello per cui si procede. Perché, se l'imputato è in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede, è condivisibile la scelta di velocizzare la trattazione del procedimento per un duplice ordine di ragioni: per evitare la scadenza dei termini della custodia cautelare e per evitare, in caso di assoluzione, di protrarre ingiustamente la detenzione. Ma se lo stato di detenzione dipende da altre cause, ad esempio da altre condanne passate in giudicato e quindi immodificabili, quale ragione giuridica, pratica e di economicità ed efficienza del sistema giudiziario può portare ad attribuire priorità assoluta al procedimento?

In secondo luogo, uguale questione di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza si pone con riguardo ai momenti processuali individuati per la sospendibilità del processo: in particolare, il termine iniziale consistente nella fissazione dell'udienza preliminare. Non appare infatti giustificabile la differenza di trattamento rispetto, ad esempio, al caso di chi abbia già assunto la qualità di imputato a quella data, con la richiesta di rinvio a giudizio, ma non abbia avuto ancora la fissazione dell'udienza preliminare. Si pensi poi, ancor di più, alla differenza di trattamento rispetto ai processi che non passano per nulla dall'udienza preliminare perché a citazione diretta in giudizio da parte del pubblico ministero. Altro elemento di problematicità, segnalato anche dall'Associazione nazionale magistrati, è che tale previsione finirà per determinare un blocco burocratico dei già lenti meccanismi giudiziari: infatti, per migliaia di processi da sospendere si dovranno impegnare risorse e personale per provvedimenti di sospensione, notifiche, udienze di smistamento e di ripresa del dibattimento, che finiranno per determinare uno stallo dei lavori giudiziari piuttosto che una loro velocizzazione. Ancora, non è comprensibile il meccanismo descritto dal comma 7 dell'emendamento, che prevede il potere del presidente del tribunale di sospendere i processi quando i reati siano prossimi alla prescrizione e le pene indultabili. Resta da comprendere come questo potere si armonizzi con il dettato dell'articolo 1, che invece prevede una sospensione immediata e per legge, senza alcuna discrezionalità del giudice. L'unica interpretazione utile possibile è che detta sospensione facoltativa riguardi anche i reati a priorità assoluta, di cui al nuovo testo dell'articolo come emendato nei termini di cui sopra, che sono richiamati (come eccezione alla sospensione) nel comma 6 della norma. Allora, signor Presidente, avremmo un sistema in base al quale molti processi sono sospesi per legge per fare spazio a processi per altri reati, considerati più gravi, ma che possono essere a loro volta sospesi se sono prossimi alla prescrizione. Tutto ciò determina il paradosso per cui sarebbe più semplice che reati prossimi alla prescrizione fossero portati all'estinzione, piuttosto che sospendere il processo, ingolfare udienze e cancellerie a tal fine, per poi riprendere il dibattimento dopo un anno, sempre ad un passo dalla prescrizione. Signor Presidente, concludo con una considerazione. Il Presidente del Consiglio, nella lettera che ha indirizzato al Senato, ha posto una questione che noi consideriamo fondata, fondata, vale a dire il rapporto tra la politica e la magistratura. Noi riteniamo, però, che tale questione abbia innestato una priorità nella priorità:

Il titolo è il seguente: «Azione penale con priorità. Il segretario dei Democratici rompe il tabù dell'obbligatorietà». Ne leggo la prima parte: «Azione penale obbligatoria, ma secondo priorità fissate dal Parlamento. È quanto si propone di fare il Partito Democratico, se vincerà le elezioni, rompendo un tabù finora considerato intoccabile».

La proposta nasce in parte dall'esperienza che ha dimostrato la volatilità dell'obbligatorietà dell'azione penale, al punto che in alcune procure della Repubblica da tempo ormai è prassi che i capi diano indicazioni ai pubblici ministeri sui reati e dunque sulle indagini da fare a cui dare la precedenza, nell'impossibilità di perseguire tutti allo stesso modo. Il primo ad introdurre questa prassi fu Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica di Torino. Dunque, in campagna elettorale avete detto le stesse cose che adesso vengono recepite

Noi abbiamo vinto le elezioni anche perché in campagna elettorale abbiamo promesso di cambiare le cose, cosa che voi non siete riusciti a fare in due anni di Governo, e di lottare contro la criminalità e l'immigrazione clandestina presenti nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi LNP e Voi state ostacolando l'approvazione di questo decreto-legge al quale seguirà poi un disegno di legge sul pacchetto sicurezza, che darà risposte concrete alla gente che vive sul nostro territorio. Noi non prendiamo in giro i nostri elettori - ed è di questo che ci stiamo occupando voi invece state ancora una volta cercando di strumentalizzare la politica per delegittimare un Governo che governerà per cinque anni. Gli elettori ci hanno votato per cambiare questo Paese

dimostrare con il suo intervento. Noi protestiamo non alla faccia di qualcuno, ma nell'interesse delle italiane e degli italiani. Questo è un momento grave e noi manifestiamo il nostro disagio, che poi è il disagio di gran parte del Paese,

Voglio ricordare alla senatrice Finocchiaro, che forse attraverso la televisione seguirà questo intervento, che con questo emendamento

Ed è per questo che chiediamo di anticipare - come disse, qualche tempo fa, perfino Piero Fassino e come scrisse il procuratore Maddalena - alcuni processi su materie incandescenti di grave allarme sociale. GARRAFFA *(PD)*. Che c'entra Berlusconi?

tant' è vero che non gradite le norme sull'impiego dei militari, sulla maggiore severità nei confronti dei clandestini, sull'accelerazione dei processi per reati di grave allarme sociale. sociale. Per quanto riguarda poi le leggi *ad personam* e le immunità, non vorrei dover ricordare che siede in quest'Aula un senatore a vita che ha usato la televisione per dire «Non ci sto» quando doveva rispondere di alcune vicende che lo riguardavano personalmente. *(Applausi dai Gruppi*

Tra lei e Macaluso, scelgo Macaluso da citare. Lei, senatore Garraffa, potrei citarla in tribunale. Dice il senatore Macaluso: «Correva in Sicilia ma era candidata al Senato in altre Regioni». Come a dire: sono qui per dare una mano e poi me ne vado. Non vorrei che la senatrice Finocchiaro se ne andasse troppo presto; vorrei che stesse in Aula a confrontarsi con noi, nel rispetto delle idee reciproche e con un contributo alla fatica della democrazia. Concludo, cari colleghi del Partito Democratico. Forse dovreste riflettere sulla vostra crisi. In questo momento ci sono più esponenti del Partito Democratico in quest'Aula che elettori del Partito Democratico in Sicilia. Questa è la realtà.

Collega Bonino, il riparto dei tempi prevede per i voti in dissenso complessivamente 10 minuti.

Ferrara).* Essere leali non vuol dire essere servi e neanche essere a busta paga.

Signori colleghi, penso che questo Senato, questa vostra maggioranza stia per scrivere una pagina PdL)*. Capisco il vostro disagio. Capisco anche la vostra insofferenza. Vedete,da noi radicali, per tutta la nostra storia, non avete mai visto cedimenti forcaioli o giustizialisti. Sulla giustizia, dal caso Tortora in poi e prima ancora, ci avete visti impegnati per la giustizia giusta, anche in situazioni impopolari, quando non additati al pubblico ludibrio. Da qui e da noi avete sentito sollevare, isolati, soli e inascoltati, il problema della cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale ridotta ad arbitrarietà dell'azione penale. Fa impressione, cari colleghi, sentirlo dire da voi oggi e non ieri e non l'altro ieri; fa impressione perché pare che ve ne siate accorti solo perché qualcuno tra voi è stato scoperto dai suoi legali... L'ha detto lui nella sua lettera! Rivendicate almeno la sua trasparenza. Lalettera è stata uno strumento inusuale, ma il Presidente del Consiglio ha voluto almeno così assumere una responsabilità chiara, non condivisibile, perché chiunque abbia a cuore la riforma della giustizia sa bene che non l'avrebbe affrontata né per decreto, né per sospensione dei processi, né l'avrebbe affrontata in questo modo, ma altre occasioni ha avuto in cinque anni passati e altre ne aveva davanti. Sicché non è un sospetto quello che circola, è la verità. Ed è per questo che mi ispira sconforto e sgomento, perché tanti anni abbiamo dedicato alla giustizia giusta, alle riforme mai attuate in questo Paese. Così non si aumentano né la sicurezza, né lo stato di diritto per i cittadini italiani. Solo per uno, ma non per i cittadini italiani.

Aggiungo che questo emendamento è un'incursione dentro lo stesso decreto che manifesta un intervento surrettizio per incidere sulla questione giustizia. La riforma della giustizia è necessaria in questo Paese, ma non si può realizzare con queste incursioni selvagge fatte a titolo personale e per i propri

Non è un buon esempio. Lo dico ai colleghi che lo hanno fatto e che sono rimasti in Aula votando anche per chi era fuori.

strada. Premetto che naturalmente dobbiamo fare tutto il possibile per garantire o almeno aumentare la sicurezza sulle strade.

Ciò che dovremmo fare, e molto più intensamente, è investire di più sull'informazione e sulla prevenzione.

a migliorare la preparazione dei neopatentati con un'esercitazione in un "centro di guida sicura". Spero veramente che l'Aula apprezzi questo emendamento e spero anche nella sua approvazione. Da una parte,

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 4.0.100, che mi appresto a illustrare, ha l'esclusivo scopo di migliorare l'efficacia delle norme contenute all'articolo 4 inerenti alle modifiche al codice della strada. Non deve sorprendere la sostanziale condivisione delle misure di pena indicate, cioè l'inasprimento delle sanzioni al codice della strada introdotte con l'articolo in parola. Molti colleghi presenti nella precedente legislatura ricorderanno infatti che la sostanza delle norme di detto articolo era stata di fatto già approvata da questa Aula e soltanto la fine anticipata della legislatura non ha consentito all'altro ramo del Parlamento di far sì che le stesse potessero effettivamente divenire leggi dello Stato. Sorprende piuttosto, ed è questo il mio appunto, come sia assolutamente assente quella cornice di riferimento che i colleghi dell'allora opposizione, oggi maggioranza, contribuirono non poco a determinare e che costituì l'elemento di successo di quei parziali provvedimenti introdotti con il decreto di anticipazione di settembre, che ancora più forza avrebbero avuto se fosse entrata in vigore la legge solo da questa Aula approvata. Cari colleghi della maggioranza, ricorderete certo con me che tutti noi insieme, appena pochi mesi fa, sostenevamo (e voi con più forza di noi) che l'inasprimento delle sanzioni, che noi allora volevamo, avrebbe avuto il risultato atteso solo se si fossero intensificati solo se si fossero intensificati i controlli effettuati sulle strade dalle Forze di polizia e se avessimo agito anche sulla prevenzione degli incidenti, a partire dalle azioni e dagli interventi concretamente possibili nei consueti luoghi di aggregazione giovanile. Fu proprio grazie al vostro contributo, con l'accoglimento di diversi emendamenti da voi proposti, che il provvedimento legislativo si arricchì di quelle misure di prevenzione e di controllo risultate, in questi pochi mesi, capaci di modificare un *trend* negativo. Oggi le riproponiamo noi a voi, non certo per un gioco delle parti, ma per un'intima convinzione che si ha e si deve avere nei confronti delle cose giuste e necessarie: norme finalizzate ad aumentare i controlli sulle strade che, come tutti noi sappiamo, sono l'unico vero deterrente ai comportamenti di guida scorretti e pericolosi. L'emendamento in proposito stabilisce che almeno l'importo derivante dall'aumento delle sanzioni previsto dalle nuove norme venga assegnato alle forze dell'ordine e destinato ad aumentare i controlli sulle strade. Al riguardo, sarebbe perfino fin troppo facile polemizzare sul fatto che, per mantenere gli impegni e le promesse fatte nella vostra campagna elettorale, per il provvedimento di copertura dell'ICI avete tolto tutte le risorse aggiuntive che noi avevamo stanziato con la finanziaria 2008, in questo e negli anni prossimi, per i controlli stradali. Date almeno, con l'accoglimento dell'emendamento, il segno della buona volontà; altrimenti, davvero i provvedimenti in approvazione saranno soltanto destinati a restare norme di carta e ad accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Lo stesso emendamento si propone anche di recuperare almeno quella parte di azioni di prevenzione richieste ai gestori e ai titolari dei locali notturni e delle discoteche, come la fornitura gratuita di etilometri prima dell'uscita dai locali, per consentire la misurazione volontaria delle proprie condizioni psicofisiche, o la predisposizione di appositi locali di decompressione o, ancora, il divieto di somministrazione di superalcolici dopo una certa ora. Sono tutti provvedimenti da voi presentati solo pochi mesi fa e da noi accolti. Infine, sempre nell'emendamento, si chiede semplicemente che venga prevista la trasmissione dei principali dati sugli incidenti stradali da parte dalle forze di polizia al Ministero dei trasporti, al fine dell'aggiornamento degli archivi previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, per dare quei presupposti minimi di conoscenza circa la localizzazione dei principali fattori di rischio sulle strade italiane. Si tratta, insomma, di norme di buon senso da voi precedentemente proposte e sostenute e per le quali sarebbe davvero incomprensibile un vostro comportamento preclusivo.

è un invito al ritiro quella soglia di sicurezza stradale che noi, invece, riteniamo debba essere elevata, vorrei dire soltanto che non si tratta di un mero incremento di sanzioni penali, anche perché si evita il giudizio di comparazione con le attenuanti e quindi vi è un effetto di dissuasione più significativo, ma vi è anche un più articolato intervento sul fermo amministrativo e sul sequestro e la confisca dei veicoli, rispetto ai quali le preoccupazioni dei presentatori degli emendamenti (come fare se si possiede una sola autovettura) possono possono essere tranquillamente affrontate decidendo di rispettare le regole del codice della strada, come avviene in ogni Paese civile. Inoltre, se mi permette di dirlo, ritengo poco riguardoso nei confronti delle forze di polizia sostenere, come abbiamo ascoltato in quest'Aula, che tali norme sono particolarmente rigorose

Presidente, volevo brevemente sottolineare ai relatori e al Governo questa ipotesi di riformulazione dell'articolo 5, che consente di colpire la concessione di alloggi a stranieri irregolari a fronte di qualsiasi tipo e genere di corrispettivo. Infatti lo scambio avviene tra alloggio e prestazione lavorativa in nero (che non sarebbe coperta dalla formulazione attuale) ovvero tra alloggio e, a volte, prestazione sessuale, piuttosto che, come avviene ordinariamente, tra alloggio e denaro. Poiché è stato introdotto il concetto di ingiusto profitto, che noi condividiamo, il testo che proponiamo serve a migliorare la formulazione dell'articolo 5 e a renderlo più efficace.

ad una pena non superiore ai due anni, possa darsi l'espulsione. Noi proponiamo di elevare questa pena a cinque anni e di raddoppiare il termine del divieto a rientrare in Italia Questo per la semplice ragione, come ormai hanno pubblicato tutti i giornali, che c'è una recrudescenza di questo tipo di criminalità degli extracomunitari e mantenere in carcere questa gente costa ben 3.500 euro al mese. Quindi, ci sarebbe un risparmio enorme e risulta molto più conveniente espellere anche chi ha commesso dei reati puniti con pena superiore a due anni,

L'integrazione dei lavoratori è una misura fondamentale per contrastare l'insicurezza, perché favorisce il contrasto delle organizzazioni e dei comportamenti criminali anche non organizzati, di singoli (quali i caporali)

i lavoratori immigrati che vengono criminalmente sfruttati con il lavoro nero; è fondamentale perché sottrae queste persone alla spinta a delinquere, cui sono maggiormente soggetti proprio i lavoratori invisibili; infine, è fondamentale perché determina lealtà nei comportamenti imprenditoriali, dal momento che spesso le imprese illegali o che sfruttano il lavoro illegalmente hanno la capacità di distorcere il mercato e le normali regole della concorrenza. Per tutte queste ragioni invitiamo ad approvare

degli irregolari sono *overstayers.* Senonché ci siamo accorti, nel passaggio tra la Commissione e l'Aula, che questa norma si pone in contrasto con il Regolamento dell'Unione europea n. 562 del 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Aggiungo che sia il Consiglio dell'Unione europea che il Parlamento europeo hanno in corso di elaborazione una proposta di regolamento recante modifica dell'istruzione consolare comune relativa agli elementi biometrici e riguardante le domande di visto. Si tratta pertanto di una materia che in questo momento è all'attenzione esclusiva dell'Unione europea, rispetto alla quale non ci possiamo certamente porre in contrasto. Sull'ordine

il termine "riconsiderare", tenendo conto che già in sede di espressione del parere sui decreti legislativi di extracomunitari e di comunitari sono state presentate proposte da parte dei relatori ai pareri di inserire esattamente la disciplina recata da questo ordine del giorno. Da ultimo,

alimenta una serie di fondi, tra cui anche quello delle vittime della criminalità mafiosa. Sarebbe opportuno esaminare nel dettaglio i contraccolpi per evitare poi squilibri nell'erogazione delle somme alle vittime della mafia;

e che intervenire immediatamente con una norma primaria salterebbe passaggi essenziali. Sono comunque disponibile, a nome del Governo, ad accogliere un ordine del giorno che spinga a tenere conto dell'istanza proveniente dal Senato.

per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Anche per quanto riguarda la contrattazione, qui si vanno a mettere risorse

Grazie

Non annoio il Senato con una questione interpretativa sul punto; considero però che, essendo in corso di realizzazione un regolamento che uniforma la disciplina per tutta l'Unione Europea, sia effettivamente opportuno rimandare, in questo quadro di organicità, a quella normazione sovranazionale.

è radicalmente diversa da quella contenuta nel decreto-legge in vigore. Nel decreto-legge in conversione si è introdotto il delitto di cessione onerosa di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante,

norma totalmente diversa. Infatti, non sarà più delitto dare alloggio oneroso allo straniero irregolare. Perché sia delitto, si richiede che ciò avvenga «al fine di trarre ingiusto profitto». gli stranieri irregolari, sfruttati da speculatori senza scrupoli, diventano parti offese e, ove lo vogliano, potranno costituirsi parte civile nel processo a carico del proprietario ingordo che abbia dato, dietro corrispettivo, un alloggio privo di requisiti minimi per assicurare una civile permanenza. L'Italia è il primo Paese che così tutelerà lo straniero clandestino dalla vessazione degli approfittatori ingordi e, nel contempo, garantirà al clandestino il diritto al risarcimento. Non posso che dichiararmi orgoglioso di essere italiano e di appartenere a questa nobile Assemblea nel momento in cui si consegna al Paese una norma di grande civiltà, degna della migliore Italia. Il mio voto è favorevole e invito l'opposizione ad un voto unanime che sottolinei con forza questo momento particolarmente solenne, espressione di massimo rigore, solidarietà e civiltà.

prego.

siano fattispecie molto serie di sfruttamento che restano fuori dall'applicazione della norma. Poiché è stato correttamente inserito il concetto dell'ingiusto profitto, se nel passaggio alla Camera questo aspetto potrà essere rivisto, la norma sarà obiettivamente perfetta. In ogni caso, il nostro voto è favorevole.

Signor Presidente, in materia di cessione di immobili avevamo presentato un emendamento più articolato che parlava di stato di bisogno, di approffittamento, di ingiusto profitto, di corrispettivo gravemente sproporzionato,

soprattutto sulla base della considerazione indiscutibilmente vera che vi sono troppi stranieri e troppi irregolari e che da questo eccesso di presenze scaturiscono conseguenze spesso anche di violenza e di illegalità, allora noi proponiamo costruttivamente un istituto che non è nuovo nel nostro Paese, il rimpatrio volontario assistito, che peraltro in Stati europei importanti ha dato risultati eccellenti sul piano dell'aumento degli allontanamenti effettivi

Kosovo. Con il rimpatrio assistito la gestione delle politiche migratorie migliora sensibilmente, proprio perché favorita dalla certezza dell'allontanamento, a sua volta resa possibile dalla collaborazione fattiva dello straniero.

per ragioni che non riesco a comprendere, si rigetta. Proponiamo di estendere il rimpatrio assistito agli irregolari e giova rilevare che il ricorso all'istituto produrrebbe nel nostro Paese un doppio beneficio, di carattere economico e di ordine pubblico e da un punto di vista politico e morale. A fronte di tante conseguenze negative, anche luttuose, secondo me non basta coprirsi la coscienza con i minuti di silenzio, bisogna operare perché siano risolti questi problemi alla radice. I rimpatri assistiti devono essere evidentemente garantiti da un fondo, che in parte già esiste e il cui costo sarebbe certamente di gran lunga inferiore ai costi che affrontiamo e che ci prepariamo ad affrontare: pensare che sono stati previsti la costituzione di nuovi centri di permanenza e l'allungamento ad un anno e mezzo della detenzione amministrativa. Andremo incontro a difficoltà insuperabili anche e soprattutto dal punto di vista economico, allora perché non accedere a questo istituto che certamente di gran lunga superiore rispetto ad ogni altro strumento? Con l'emendamento in esame vogliamo suggerire e proponiamo l'adozione di uno strumento che, se adottato, farà risparmiare ai contribuenti italiani e in maniera indolore determinerà un abbassamento sensibile del numero degli irregolari. È previsto, ovviamente, che l'irregolare assistito per il rientro nel suo Paese che dovesse rientrare prima del tempo previsto dalla legge meriterà allora certamente una pena detentiva. abbassiamo i termini per la possibilità del rientro per coloro i quali volessero liberamente e spontaneamente accedere a questa procedura di allontanamento. e sterile i muscoli, aumentare le pene, organizzare nuovi centri di permanenza, affrontare - non so ancora in che modo - il problema drammatico delle carceri italiane, che hanno già raggiunto quota 60.000 e che con questo decreto e con altre norme che la maggioranza si accinge a varare

innanzi tutto ringrazio il Governo per aver accolto l'ordine del giorno nel quale chiedo di superare l'equiparazione esistente

sociale. Mi chiedo, vi chiedo colleghi senatori e chiedo al Governo: è corretta, è giusta, è giustificata questa equiparazione? Prima

perché credo di aver fatto bene a denunciare, peraltro con la pacatezza di sempre, un fenomeno antipatico. Quando i colleghi sono usciti dall'Aula,

ragione io pianista non lo sono mai stato, ancorché sono finito sul «Corriere della Sera», su «Striscia la notizia», eccetera. Il senatore Garraffa, probabilmente faceva erroneamente riferimento a quelle vicende, ma il tribunale e quindi i giudici, che tanto giustamente vengono difesi in quest'Aula,

L'intervento di oggi, viceversa, è a difesa dell'onorabilità del sottoscritto; però la Presidenza è informata di questo. La prossima volta, dovesse accadere un fatto del genere, prego la Presidenza di correggere immediatamente, così come chiedo le scuse

Grazie